L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione,

la partecipazione italiana alle missioni internazionali e agli interventi di cooperazione e sostegno nei processi di pace e stabilizzazione. Il provvedimento, a differenza del passato, assicura una copertura degli interventi sull'intero anno solare di riferimento.

agisce per la stabilizzazione delle aree critiche e il superamento degli scenari conflittuali. L'approccio dell'Italia si connota, peraltro, storicamente per la capacità di coniugare la dimensione militare con quella civile, nell'ottica di garantire una duratura stabilizzazione delle principali aree d'intervento. In questa direzione devono intendersi rivolti gli interventi e le iniziative in ambito umanitario che vanno ad affiancarsi sempre alle missioni internazionali in senso stretto. Sottolineo l'espressione «affiancarsi sempre alle nostre missioni internazionali» perché - come abbiamo avuto modo di vedere anche nel serio dibattito che le due Commissioni hanno condotto su questa materia

e della cattiveria delle azioni di Daesh e del fondamentalismo islamico. Lascio ovviamente al collega Vattuone l'illustrazione del Capo I di questo provvedimento che riguarda le missioni militari. Per i profili concernenti gli affari esteri, di cui al Capo II del decreto-legge, sottolineo in primo luogo che la spessa complessiva per le misure di cooperazione e stabilizzazione ammonta a 260 milioni di euro. Nel dettaglio, per iniziative di cooperazione allo sviluppo, previste dall'articolo 8, sono autorizzate risorse per 90 milioni di euro, finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e al sostegno alla ricostruzione civile in una serie di Paesi: Afghanistan, Burkina Faso, Etiopia, Repubblica Centrafricana, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Palestina, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen e nei Paesi a essi limitrofi, per la necessaria assistenza ai rifugiati. Si tratta di fondi destinati a integrare gli stanziamenti già disposti dalla legge sulla cooperazione allo sviluppo. A tal riguardo A tal riguardo ricordo che la legge di stabilità per il 2016 aveva disposto stanziamenti collegati a interventi di cooperazione allo sviluppo per 1,199 miliardi di euro, con riferimento allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, e per ulteriori 380 milioni di euro con riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'economia Con riferimento all'Afghanistan, i finanziamenti danno seguito agli impegni assunti dall'Italia nelle conferenze di Bonn e di Tokyo, e sono destinati a interventi prioritari per il sostegno alle finanze pubbliche e lo sviluppo socio-economico della popolazione, oltre che per programmi di sviluppo rurale, di *governance*, di salvaguardia dei diritti delle donne e di tutela del patrimonio culturale. le misure sono indirizzate prevalentemente al settore dello sviluppo rurale, con particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili, mentre in Myanmar al rafforzamento delle capacità delle istituzioni istituzioni locali e al sostegno del patrimonio culturale. Gli interventi in Iraq sono finalizzati a misure umanitarie, in particolare per gli sfollati interni. L'impegno è indirizzato, in particolare, a favore delle Agenzie ONU presenti nell'area (dall'Unicef all'Alto commissariato per i rifugiati), col supporto delle università e della cooperazione decentrata italiane. In Siria e nei Paesi limitrofi le iniziative sono rivolte ai settori dell'agricoltura e della sicurezza alimentare, oltre che al sostegno alle comunità ospitanti, e a sostenere la partecipazione italiana ai fondi fiduciari regionali per la crisi, fra cui il Fondo europeo, che vede l'Italia fra i cofondatori, e che nel 2015 ha gestito finanziamenti per quasi 500 milioni di euro. Altri interventi qualificanti sono destinati, tra l'altro, ai territori palestinesi (in particolare per la ricostruzione di Gaza), alla Libia (per iniziative nei settori agricolo, di sviluppo rurale, sanitario e dell'istruzione), alla Somalia (per il sostegno ai servizi sanitari di base), allo Yemen allo Yemen (per fronteggiare le conseguenze della guerra civile), al Sudan (per il consolidamento del processo di pace nell'area orientale e per l'attività umanitaria in Darfur) e al Sud Sudan (per fronteggiare l'emergenza in atto e per il rafforzamento delle condizioni di sicurezza alimentare). Particolare attenzione viene data alla diffusione pubblica dei risultati ottenuti attraverso questa attività, che sono pubblicati sul sito Internet istituzionale del Ministero, Una spesa di 1,7 miliardi di euro è poi destinata alla realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, da realizzarsi principalmente in Afghanistan, Somalia, Siria, Libia, Colombia, Iraq e a Gaza. Relativamente alle misure di sostegno ai processi di ricostruzione, di pace e di stabilizzazione, l'articolo 9 autorizza una spesa complessiva per circa 168 milioni di euro. Di questi, 6 milioni sono destinati a interventi per sostenere i processi di pace, di stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza in Paesi come l'Afghanistan, l'Iraq, la Libia, la Siria, la Tunisia e nei Paesi dell'Africa subsahariana, dell'America latina e caraibica. Un impegno specifico è destinato a sostenere la riconciliazione nazionale e la transizione democratica in Libia e per la stabilizzazione in Iraq e Siria e a beneficio dell'economia tunisina gravemente colpita dagli attentati del 2015. 2,1 milioni di euro sono destinati al finanziamento di fondi fiduciari (come quelli della NATO, per il rafforzamento delle istituzioni e degli enti di difesa di Paesi *partner*, e dell'ONU, per la soluzione delle crisi libica e siriana), e di alcuni programmi delle organizzazioni internazionali (fra cui il programma UNDP in Libia), oltre che a beneficio dell'Unione per il Mediterraneo e del Tribunale speciale ONU per il Libano.

in esame finanzia, inoltre, interventi operativi di emergenza e sicurezza per la tutela dei cittadini e delle strutture della rete diplomatica in aree di crisi, per un totale di 27,5 milioni di euro, riferendosi, in particolare, ad aree come l'Afghanistan, l'Egitto, i territori palestinesi, l'Arabia Saudita e la Somalia. L'articolo 9 del provvedimento disciplina il trattamento per il personale del Ministero inviato in missione nelle sedi a rischio, mentre l'articolo 10 stabilisce il regime di interventi e contiene alcune disposizioni derogatorie alle normative vigenti in materia. Di interesse appare soprattutto il comma 3 dell'articolo volto a modificare un articolo della nuova legge sulla cooperazione allo sviluppo (legge 11 agosto 2014, n. 125), al fine di istituire uno specifico conto di tesoreria cui far affluire le risorse destinate agli interventi di cooperazione distinto da quello destinato alle spese di funzionamento dell'Agenzia, senza peraltro nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- che introduce il tema del nostro intervento di cooperazione, di sostegno allo sviluppo e assistenza alle popolazioni, ai processi di democratizzazione di democratizzazione ed evolutivi in atto in varie parti del mondo, ovviamente giovandosi delle missioni militari quale supporto indispensabile alla politica È evidente che, se si decontestualizzano

In questo senso, la politica estera viene prima della politica militare, ma la politica militare diventa parte integrante di una politica estera per la pace, la stabilizzazione, la multilateralità e l'affermazione delle organizzazioni internazionali. *(Applausi

il decreto‑legge in esame, che il Parlamento si accinge a convertire, affronta il tema delle missioni internazionali riferite al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016. Il collega Sangalli ha compiuto una disamina dello scenario internazionale che continua a presentare molteplici elementi di instabilità; una condizione, purtroppo che, si traduce per l'Italia, come per la comunità internazionale in cui siamo inseriti, in un costante rischio per la nostra sicurezza. I gravi attentati che si sono verificati in Europa nei mesi passati hanno potuto confermare il legame tra i conflitti in atto nelle regioni che circondano il Vecchio continente e la sicurezza all'interno dei nostri Stati. hanno confermato la capacità operativa dei gruppi terroristici che sanno operare in contesti bellici veri e propri e che riescono a infiltrarsi nelle nostre città. Hanno altresì confermato il grave rischio rappresentato dai cosiddetti cosiddetti *foreign fighter*, che hanno acquisito conoscenze e capacità militari combattendo nelle guerre civili e che possono ora utilizzare tali competenze per finalità terroristiche. Questo insieme di fattori rende evidente l'importanza, oggi più di ieri, dell'azione portata avanti dalle nostre Forze armate e di polizia; azione che si svolge - come è ben noto - tanto nei teatri di crisi all'estero quanto sul territorio nazionale e nelle acque attorno ad esso. In questo quadro, nel decreto-legge missioni si evidenzia da subito un particolare sforzo verso il contrasto al terrorismo, anche e soprattutto in relazione all'area mediterranea. La politica di difesa e sicurezza rappresenta sicuramente uno dei fattori maggiormente condivisi in ambito internazionale e uno degli ambiti in cui da tempo era stato definito l'obiettivo di una politica comune europea maggiormente integrata, politica comune che, per quanto insufficiente, ha dato un contributo significativo, insieme all'altro pilastro rappresentato dalla NATO, a mantenere il sistema di *governance* globale. L'Unione europea ha svolto nell'ultimo decennio un ruolo crescente nella gestione delle crisi in generale, sia a livello regionale che globale. Con la creazione e la successiva espansione della politica europea di sicurezza e difesa, ora denominata "politica di sicurezza e difesa comune", l'Unione europea ha acquisito una serie di strumenti operativi e istituzionali per la gestione delle crisi, ancora insufficienti, certo, ma con una prospettiva assolutamente indispensabile per la gestione delle crisi. del Piano strategico per la sicurezza europea, che può rappresentare senz'altro un capitolo di rilancio dell'Unione europea. Viceversa, un'Unione europea avviata verso il declino del suo progetto cesserebbe di essere un attore internazionale di rilievo e la nostra influenza negli equilibri mondiali, nelle istituzioni multilaterali e nei grandi negoziati internazionali si ridurrebbe al minimo. Invece di un *partner*, gli Stati Uniti avrebbero nell'Europa un problema la solidità dell'Occidente, così come la sua capacità di esercitare una *leadership* si incrinerebbe. Perderebbe forza e vigore la stessa idea che le relazioni internazionali debbano essere completate da istituzioni multilaterali, da alleanze, regole e pratiche condivise, a vantaggio di una visione del mondo basata su unilateralismi e nazionalismi anacronistici. Questo è particolarmente evidente nei Balcani, per fare un esempio. Per i Paesi di quest'area l'Unione europea è ormai diventata il principale punto di riferimento politico-economico. Credo che nessuno possa avere dubbi sul fatto che solo attraverso la collocazione nelle organizzazioni internazionali - come diceva bene il collega Sangalli a conclusione del suo intervento

per essere il più vicino storicamente agli interessi e alle priorità del nostro Paese. L'Italia ha operato, dall'inizio di questa legislatura, affinché l'area del Mediterraneo divenisse una priorità per l'Unione europea e per la NATO e, con Mare nostrum, ha saputo assumere un ruolo trainante nell'agenda politica internazionale dell'Unione europea. Il risultato è oggi confermato dall'impegno comune nel contrasto ai traffici di esseri umani nel Mediterraneo centrale, estendendo di un anno la missione EUNAVFOR Med, cui si aggiungono altre due funzioni, una di addestramento della guardia costiera libica in acque internazionali e l'altra di contributo al controllo dell'embargo, che continua a essere violato. Ci sono poi l'accordo per il *migration compact*, che rappresenta la strategia di partenariato con i Paesi di origine e di transito dei flussi migratori, e la risposta positiva degli Stati Uniti alla richiesta dell'Italia di rafforzare il fianco Sud della NATO, realizzando tra l'altro quel coordinamento strategico tra NATO e Unione europea che l'Italia ha proposto e sostenuto con vigore negli ultimi mesi. Entrando nel merito, per quanto attiene agli aspetti di stretta competenza della Difesa e per la parte riferita alle Forze armate, il provvedimento è strutturato secondo le consuete modalità, suddividendo le missioni in tre articoli sulla base della dislocazione continentale dei contingenti (Europa, Asia e Africa). È confermata la disciplina costantemente reiterata dai provvedimenti legislativi di proroga delle missioni con riguardo al personale, alla materia penale e a quella contabile. La consistenza media annuale del personale impiegato è pari a circa 5.938 unità, con un incremento di circa 245 unità rispetto alla media registrata nell'ultimo trimestre dell'anno 2015, per un impegno di spesa nella difesa di circa 1,017 miliardi. In particolare, è rafforzata la partecipazione alle attività della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh (da 750 a 978 unità), prevedendo, a decorrere dal 1° aprile 2016, un dispositivo di *personnel recovery* per attività di ricerca, individuazione e recupero del personale rimasto isolato in ambiente ostile, composto di una ulteriore aliquota di personale (137 unità) e dei relativi assetti aeromobili. Inoltre, su richiesta della coalizione internazionale e d'intesa col Governo iracheno, l'Italia - come è noto - si è resa disponibile a garantire la protezione dell'area della grande diga di Mosul, opera strategica per tutta la regione, dove sta avviandosi il progetto per il suo consolidamento, per scongiurarne il crollo e i conseguenti immensi danni che questo provocherebbe. Per quest'ultimo impegno, sono state compiute le attività preliminari di ricognizione dei luoghi. Oggi, come previsto nel decreto-legge sulle missioni, con l'emendamento proposto dal Governo, già approvato dalle Commissioni 3a e 4a riunite, in aderenza con gli sviluppi complessivi del progetto, si procede all'effettivo invio di personale nel teatro operativo scaglionato nel tempo, per un totale di circa 500 unità entro il mese di ottobre 2016.

cui abbiamo discusso anche in Commissione, è essenziale per la sicurezza marittima nel Mediterraneo; è confermata la consistenza media del personale impiegato (753 unità) che, con le unità impegnate, garantisce la sicurezza delle fonti energetiche strategiche, dei transiti commerciali e delle attività di pesca.

al potenziamento dei dispositivi dell'Alleanza atlantica, in ossequio al principio di solidarietà fra alleati in vari teatri. Si tratta di nuove disposizioni che nel dettaglio sono: l'operazione della NATO Active fence consiste nello schieramento di batterie antimissile a difesa dei confini sudorientali dell'Alleanza. Si tratta di contribuire per sei mesi

Vi sono poi misure di rassicurazione nella regione sudorientale con il potenziamento del dispositivo per la sorveglianza dello spazio aereo dei Paesi membri dell'Europa orientale e dell'area sudorientale dell'Alleanza, e quindi ai confini dell'area NATO. In questo caso vi sono le autorizzazioni per rendere disponibile un velivolo da rifornimento che potrà operare a favore della componente alleata di aerei radar, impegnati a garantire la sorveglianza dello spazio aereo. Vi è poi un potenziamento del dispositivo per la sorveglianza navale dell'area Sud dell'Alleanza, dove l'Italia partecipa con un cacciamine. È prevista la proroga, fino al 31 dicembre 2016, dell'impiego di 1.500 unità di personale delle Forze armate per le esigenze di sicurezza

e Africa. Gli articoli 5, 6 e 7 recano le consuete disposizioni in materia di personale, penale e contabile. Si rilevano, tuttavia, due interventi innovativi dell'ordinamento. Per quanto attiene le disposizioni penali, vengono introdotte alcune modifiche all'articolo 10 del codice di procedura penale. In materia contabile viene introdotto, all'interno del codice dell'ordinamento militare, un nuovo articolo in materia di contratti di assicurazione e trasporto. Vi sono stati alcuni emendamenti approvati in Commissione. Io e il collega Sangalli, in qualità di relatori,

preposta al perseguimento delle funzioni di interesse pubblico secondo le disposizioni legislative vigenti, nonché quelle di concorso alla formazione in materia di emergenze e di protezione civile.

probabilmente perché l'obbligo di costituzione della Fondazione, oggi già previsto, non è assistito da un termine perentorio né da rimedi sostitutivi. La norma, pertanto, non introduce nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto le attività della Fondazione, come oggi delineato dalla normativa vigente, saranno finanziate mediante la contribuzione pubblica a carico delle amministrazioni interessate (sono la Difesa e l'Economia), attraverso il ricorso alla convenzione già contenuta e nei limiti e nelle norme attualmente previste. Anche per quanto attiene al personale, l'emendamento non introduce nuovi o ulteriori oneri, in quanto riproduce la formulazione vigente. Da ultimo, figurano le norme sulla copertura finanziaria e sull'entrata in vigore. Concludo formulando un ringraziamento sincero alle nostre Forze armate per l'impegno dimostrato, con serietà e professionalità riconosciuta a tutti i livelli, ribadendo ancora una volta che il nostro Paese vanta un impegno di lungo periodo, rimanendo tra i più importanti Paesi contributori, sia in termini di personale impiegato sia per quanto concerne il contributo finanziario. nella realtà complessa e travagliata di oggi, le missioni internazionali sono uno degli strumenti privilegiati per affrontare le crisi complesse e attuare una politica internazionale adeguata alle nuove difficoltà e crisi. Il nostro impegno è sostenuto da principi base che orientano e sovrintendono alla nostra politica estera e di sicurezza, che seguiamo da molti anni e che discendono dal secondo periodo dell'articolo 11 della nostra Costituzione. Mi riferisco alla nostra scelta per la gestione multilaterale delle crisi e per conferire stabilità, continuità e capacità di programmazione all'azione della comunità internazionale a favore della stabilità e dello sviluppo pacifico, in un contesto di adesione al sistema di relazioni e istituzioni basato sulle Nazioni Unite e le altre organizzazioni cui apparteniamo in conformità al diritto internazionale.

alcune vanno avanti praticamente da oltre un decennio. Non si capisce perché si insista in questo tipo di missioni militari che, evidentemente, non hanno portato ad alcun risultato, se c'è bisogno di continuare

ad esempio, all'articolo 9, che dovrebbe occuparsi del sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e stabilizzazione. È stato osservato da diverse associazioni che si occupano di diritti umani che, proprio al comma 3 dell'articolo al comma 3 dell'articolo 9, nel quadro dell'impegno finanziario della comunità internazionale per l'Afghanistan, si stanziano 120 milioni di euro a sostegno delle forze di sicurezza afgane, comprese le forze di polizia; analogo provvedimento con una somma diversa è previsto per le forze di polizia somale. somale. Vorrei ricordare che, a detta di più organizzazioni che si occupano di diritti umani e operano in campo internazionale, sia la polizia afgana che la polizia somala sono state segnalate alle Nazioni Unite come forze che utilizzano i bambini soldato. Non parliamo poi di tutta un'altra serie di comportamenti molto discutibili messi in atto dalle stesse forze di polizia che noi insistiamo a voler foraggiare, praticamente determinando, con il nostro contributo, il perpetuarsi di certe situazioni e l'utilizzo di bambini soldato che, finora - vorrei dirlo - nessun componente delle Forze armate o del Ministero della difesa è riuscito a smentire. Quindi, credo che vada data fiducia alle segnalazioni che ci vengono fatte da organizzazioni per i diritti umani. Per quanto riguarda la parte più squisitamente militare delle missioni, c'è praticamente ben poco di nuovo da segnalare, salvo il fatto che la situazione internazionale e i problemi da essa derivati continuano a essere sempre gli stessi. Non vedo alcun impegno da parte del nostro e di altri Governi che partecipano a queste missioni militari, per cercare veramente una svolta una svolta nelle situazioni di conflitto in cui stiamo intervenendo; una svolta che probabilmente non c'è perché nessuno la vuole. vuole. Tutto sommato, le missioni militari all'estero sono ormai diventate una *routine* nell'attività delle nostre Forze armate,

l'impiego di determinate Forze armate che altrimenti rimarrebbero inutilizzate e la spesa di notevoli risorse; soldi che poi vengono spesso utilizzati anche in maniera distorta, non proprio proprio per lo scopo per cui sono stati stanziati, ovvero per svolgere missioni militari all'estero, ma semplicemente per aumentare la disponibilità e la capacità di spesa dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Marina, che hanno hanno intrecci di interessi ormai consolidati con l'industria bellica italiana e tutto il sistema delle esportazioni delle nostre armi nel mondo, che, anziché andare a risolvere i problemi

*(PD)*. Signora Presidente, i due distinti provvedimenti di proroga delle missioni internazionali approvati nel 2015 già avevano registrato un diverso posizionamento del nostro sistema di sicurezza e difesa per adeguarlo alle nuove minacce e all'emergere di inediti e urgenti scenari di crisi. Ciò in conseguenza delle priorità emerse a seguito dei tragici fatti di Parigi, prova di un salto di qualità nella capacità di minaccia nel gruppo del cosiddetto Stato Islamico inoltre in ragione dell'opportunità di aumentare la funzione di sorveglianza e controllo nel bacino del Mediterraneo quale conseguenza della stessa emergenza migranti. È in questo quadro che, accanto agli impegni che da anni caratterizzano la nostra posizione internazionale - penso ad esempio alla presenza nei Balcani, alla missione UNIFIL nel Libano o all'Afghanistan si sono aggiunti gli impegni nella coalizione contro l'ISIS e la stessa missione EUNAVFOR Med. Il profilo della nostra azione esterna, della nostra proiezione nello scenario internazionale, nel decreto-legge di proroga delle missioni 2016, questo orientamento, segnandolo con più nettezza. risponde alla necessità di dare continuità alle azioni intraprese per il mantenimento della pace sul piano nazionale, continuità che oggi è ancora più necessaria perché i contesti quali il Libano o l'Afghanistan subiscono sistematicamente le ripercussioni dell'instabilità prodotta nell'area della regione siro-irachena e contemporaneamente della diffusione dell'estremismo jihadista. Gli stessi rapporti, poi, che descrivono la situazione in cui si trova ad operare la missione UNIFIL, dopo una prima fase in cui si era registrata una relativa tranquillità nell'area della cosiddetta *blue line*, registrano il fatto che che la stessa area libanese sta subendo il contagio del conflitto in Siria con un massiccio arrivo di profughi dalle zone di guerra ed un deciso aumento delle ostilità che ha coinvolto anche le stesse truppe di Assad sul territorio libanese. È noto ancora che anche in Afghanistan, negli ultimi mesi, i talebani hanno intensificato i rapporti con la Rete Haqqani e con Al Qaeda che, seppur ridimensionata, ha un'attiva presenza nella regione. il provvedimento al nostro esame definisce nuovi impegni, come quello relativo alla protezione della diga di Mosul o ancora l'onere assunto in ambito NATO a protezione dello spazio aereo turco dal rischio di sconfinamenti provenienti dalla Siria. Questo insieme di impegni esplicita perciò la piena partecipazione del nostro Paese nell'evoluzione dello sforzo della comunità internazionale e contemporaneamente precisa la definizione della nostra stessa collocazione nello scacchiere internazionale, tenuto conto di quelle situazioni che non possono non essere condivise nei fatti. Ciò che risulta importante, e che credo vada posto all'attenzione della nostra discussione, sono anche quelle priorità che trovano riscontro nell'interesse complessivo della comunità internazionale e che appartengono all'Italia in primo luogo, soprattutto sul fronte della nostra forte caratterizzazione nel bacino del Mediterraneo dove, com'è noto, l'Italia dalla fine del 2013 con la missione Mare nostrum si è assunta oneri e responsabilità per far fronte al massiccio aumento dei flussi migratori. In questo quadro, la missione EUNAVFOR Med è li a dimostrare, io credo, come l'azione politica diretta, volta a portare il Mediterraneo al centro dell'agenda globale, abbia dato, o almeno inizi a dare, i primi risultati.

alla richiesta dell'Italia di rafforzare il fianco Sud della NATO con un nuovo disegno strategico che vada oltre la risposta emergenziale del soccorso dei migranti, sono il frutto della nostra decisa azione politica. Il provvedimento, quindi, disegna il profilo di un Paese saldamente incardinato nella comunità internazionale, che si è via via dimostrato in grado di influire anche negli ambiti di codecisione riuscendo a far emergere nell'agenda della comunità internazionale i profili più vicini alle nostre priorità. In ogni caso, signora Presidente, la stessa vicenda collegata alla Brexit pone oggi con forza l'esigenza di rilanciare nell'ambito dell'Unione, insieme ad un ripensamento del progetto europeo, anche la prospettiva di una di una politica estera e di difesa comune, al fine di consentire all'Europa di svolgere quel ruolo fondamentale di protagonista nello scenario internazionale, su un piano di unità d'intenti, di valori e di politiche condivise, necessari per affrontare le dinamiche di un mondo in profondo cambiamento, e in difetto del quale le Nazioni europee difficilmente riusciranno a evitare l'irrilevanza e il declino. La storia dell'unificazione europea dimostra, ancora, dalle origini in poi, che i progressi verso una maggiore integrazione sono stati compiuti quasi sempre sotto la spinta di eventi esterni, a volte drammatici, come è stato per il rilancio della difesa comune dopo le guerre nella ex Jugoslavia. È nostro compito, quindi, esprimere una capacità politica che faccia sì che l'Unione europea sia in grado di ridefinire una propria, concreta identità, non più percepita come distante, legata magari alla sola dimensione degli interessi finanziari dei Paesi o del Paese più forte. Si tratta, invero, di disegnare obiettivi di lungo periodo, che siano capaci di esprimere una nuova visione, in grado di rilanciare scelte politiche ed economiche condivise, di lungo periodo appunto, per una nuova stagione di crescita e di sviluppo sociale*. (Applausi

vorrei fare una premessa. Come Lega Nord, nell'affrontare queste tematiche, siamo stati da sempre estremamente responsabili, anche perché, la politica estera di uno Stato proietta la sua immagine e la sua credibilità verso l'esterno, si possa essere di schieramenti contrapposti, la massima serietà va posta sui temi che devono essere affrontati. Così è sempre stato e così sarà,

Intanto vorremmo sottolineare una grave responsabilità comportamentale del Governo: continuiamo a discutere di proroghe di missioni in essere, ma aspettavamo questo provvedimento a Capodanno dell'anno scorso e non è arrivato. Questo significa che migliaia di marinai, piloti e soldati hanno operato finora scoperti di protezione giuridica. Ci siamo chiesti per quale motivo vi sia stata questa negligenza da parte del Governo abbiamo provato noi a capire le motivazioni di questo ritardo I casi sono due, forse tre. O il Governo ha atteso che si chiarissero due posizioni internazionali, quella dell'Iraq e quella della Libia, magari per inserire in questo provvedimento eventuali nuovi impegni,

terza ipotesi - che non è da scartare a priori - è che il Governo abbia atteso fino adesso pensando ad una

competenti per quanto riguardava la ripartizione dei soldati e delle risorse tra le varie operazioni già autorizzate nel corso dell'anno. Una delle tre. Poi vi è un giallo, che abbiamo evidenziato scrutando la cronologia: il decreto-legge viene approvato in Consiglio dei ministri il 29 aprile scorso e siamo in profondo ritardo, però passano tre settimane prima che il provvedimento venga pubblicato in *Gazzetta

lo sfruttamento e di iniziare la vera lotta al traffico di esseri umani. Questo è il fine della missione. Noi abbiamo sentito i marinai che partecipano alla missione e sono a

fungono da navi passeggeri per raccogliere e convogliare nei nostri centri d'accoglienza chiunque venga trovato in difficoltà in mare. Non si critica l'operazione di soccorso, ma il fatto che sono state destinate risorse, mezzi e strutture navali ad un fine che non era questo.

Notiamo, per dichiarazioni di organismi internazionali quali il segretariato di Frontex, che nelle casse dei terroristi sono finiti più di 5 miliardi

ad associazioni legate ad Al Quaeda, all'ISIS, a Daesh. Credendo di aiutare poveri cristi, noi abbiamo alimentato

inumani nel fare un ragionamento razionale. Chi sono queste persone che vengono aiutate in mare? Non sono poveracci. I poveracci rimangono nei loro Paesi, nelle capanne di fango, a morire di fame esattamente come facevamo prima. Infatti, chi arriva

Queste persone alimentano le casse del sistema terroristico che minaccia

Renzi ha avuto dei contatti recentissimi con le autorità russe. Renzi, il Presidente del Consiglio italiano, ha capito gli interessi energetici italiani e delle aziende italiane sono penalizzati in modo enorme dalle sanzioni antirusse e che non si sarebbe potuto continuare su questa strada.

sede che illustrerà al Consiglio europeo la possibilità di chiudere con le sanzioni o di trovare vie alternative alle sanzioni nei confronti della Russia.

di sovranità serba può essere riconosciuto internazionalmente, anche se il mio collega Stucchi oggi ha dichiarato, a nome della Lega, che noi non lo riconosciamo perché, se riconosciamo ogni Paese che si autoproclama

Oggi potrebbe leggersi come un'operazione intelligente, in quanto l'attuale Governo egiziano è impegnato nella lotta antiterrorismo, come lo sono tante altre forze, anche perché, confinando con la Libia,

a Morsi ad al-Sisi. E se domani, con una prossima elezione, ritornassero a governare - con Morsi o con un altro Presidente - i Fratelli Musulmani?

Ebbene, si sta pensando di consentire agli armatori di utilizzare dei *contractor,* cosicché chi porta un carico, e deve difenderlo in un'area in cui ci sono anche rischi di pirateria,

anni orsono. Ebbene, dovevamo pensare noi alla sicurezza, a recintare i cantieri in quelle aree, a mettere un sistema di polizia,

Grazie

tuttavia, poco coerente il fatto che i guadagni vadano alla società Trevi mentre i costi siano del popolo italiano.

un'autorizzazione all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ad assumere 60 dei 120 tecnici dell'area tecnico-operativa, in deroga alla legislazione vigente. di più. I dirigenti generali (e anche quelli di area non generale) possono ottenere l'incarico per conferimento.

e si dice che: «non si rinvengono adeguate professionalità» e pertanto si accede a procedure atipiche. Per questi motivi, che riteniamo molto pregnanti e non frivoli, vorremmo

della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. È evidente che abbiamo votato tanti decreti-legge di questo tipo e spero davvero che questa sia l'ultima volta che lo facciamo. Quando la legge quadro sulle missioni terminerà il suo percorso parlamentare avremo la possibilità,

La centralità del tema è evidente a tutti dopo la tragedia avvenuta in Francia lo scorso anno, che ha posto al centro del dibattito politico la necessità della difesa e di una strategia internazionale a contrasto dell'emergere

Tra i rilevanti contenuti del decreto-legge in esame, sottolineo l'importante proroga di missioni già attive allo stato attuale in territorio sia europeo, che extraeuropeo.

proroga per l'intero anno una serie di missioni già attive in territorio africano, mentre l'articolo 4 prevede le autorizzazioni di spesa relative a ulteriori esigenze connesse alle missioni internazionali, tra cui la stipulazione di contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione delle Forze armate. È importante sottolineare che, al fine di tutelare le esigenze di sicurezza relative al territorio italiano, il provvedimento in esame proroga per tutto l'anno l'impiego di un contingente di ulteriori 1.500 unità, rispetto alle 4.800 unità di personale già impiegate l'anno scorso, per le esigenze di sicurezza connesse al Giubileo straordinario della misericordia e ad alcune specifiche aree del territorio nazionale, impiego già autorizzato fino al 30 giugno 2016. Inoltre, dal 9 maggio al 31 dicembre è incrementato di 750 unità il contingente già utilizzato, limitatamente ai servizi di vigilanza e a siti ed obiettivi sensibili, nella misura di 4.800 unità.

ai processi di ricostruzione e per la partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. La sicurezza è certamente un valore per tutti noi e per tutti i nostri cittadini e oggi lo è ancor di più, dopo i tragici fatti di Parigi. Recentemente abbiamo sentito, dentro e fuori i palazzi istituzionali, interventi del tipo: «Richiamiamo i nostri soldati, perché abbiamo bisogno di difenderci all'interno del nostro Paese». Tuttavia non c'è posizione o atteggiamento più anacronistico di questo. Paesi storicamente neutrali, come il Giappone, la Svezia e la Finlandia, dove l'opinione pubblica è ancora ampiamente favorevole alla neutralità, hanno avviato revisioni dei propri ordinamenti o partecipano attivamente alle missioni internazionali. Oggi l'esigenza di sicurezza richiede di uscire dai propri confini, anche perché la guerra ha assunto caratteristiche diverse da quelle tradizionali. Si sente spesso parlare di guerra asimmetrica o ibrida, vengono usati i civili e si ricorre al terrorismo, alla guerriglia, alla guerra informatica e soprattutto alla propaganda. Insomma, i metodi dei conflitti e gli scenari diventano globali e ciò richiede una prevenzione a 360 gradi. prevenzione e gestione dei post-conflitti, oltre alla capacità di tenere in piedi una macchina militare efficiente. Ovviamente, ciò implica che si abbia il coraggio anche di dire no a facili demagogie e di riconoscere il valore, per l'Italia, della grande professionalità e dell'equilibrio con cui le nostre Forze armate sono presenti nei vari scenari mondiali. Noi abbiamo la responsabilità di spiegare ai nostri cittadini che le spese per la difesa sono investimenti e, al tempo stesso, che la forza o l'intervento armato militare, senza una forte identità nazionale ed europea, non è sufficiente a garantire la sicurezza di un popolo. Il ruolo che l'Italia gioca nel recupero di questa identità è fondamentale, senza dimenticare l'apprezzamento che i nostri soldati ricevono all'estero ogni volta che sono impegnati in operazioni internazionali volte al mantenimento o alla stabilizzazione dei processi di pace. Non possiamo rinunciare a sostenere la speranza di pace e di un futuro migliore rappresentato dai volti dei nostri ragazzi in missione. Dobbiamo sostenere unitamente i loro sacrifici e il loro spirito di servizio, mettendo da parte contrapposizioni e personalismi, in quanto nei loro sacrifici

Signora Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame interviene, come di consueto, in materia di politica estera e di difesa. Sarà forse l'ultima volta che voteremo un decreto-legge di rifinanziamento delle missioni, essendo in dirittura d'arrivo alla Camera la legge quadro, già approvata in Senato qualche mese fa, che supererà la desueta disciplina della decretazione d'urgenza in materia. Forza Italia, com'è noto, ha sempre votato questi provvedimenti, a prescindere dalle responsabilità di Governo, rivendicando con orgoglio l'apprezzamento e l'alta stima verso le nostre Forze armate, che si distinguono nei vari scenari ove operano per impegno e professionalità unanimemente apprezzate. In questa occasione, però, il nostro approccio rimane fortemente critico, poiché nel decreto-legge in esame, a parte le necessarie proroghe alle tante missioni cui l'Italia partecipa, si perpetuano situazioni che nulla hanno a che vedere con la sicurezza del Paese e molto con la stucchevole demagogia del Governo, che continua a finanziare missioni nate con obiettivi di sicurezza e proseguite con altre finalità. In tal senso la missione EUNAVFOR Med, per la quale risultano stanziati quasi 70 milioni di euro, nata per combattere e smantellare il traffico di esseri umani nel Mediterraneo centro-meridionale, si è trasformata, dopo la prima fase di raccolta di informazioni di *intelligence* e qualche arresto di scafisti, in una sorta di Mare nostrum 2, tradendo le ragioni per cui era stata costituita, col rischio non tanto larvato di mantenere intatto questo baraccone dell'immigrazione clandestina, per la gioia criminale di quanti in Libia, ma anche in Italia, dal fenomeno migratorio traggono benefici economici e politici. I dubbi, pertanto, che avevamo evidenziato a suo tempo, pur avendo espresso un voto positivo, si sono rivelati in tutta la loro evidenza. Solo la prima fase poteva essere esperita con un certo successo, ma di smantellare il traffico dei migranti neanche a parlarne. In questi giorni, inoltre, è stato attribuito alla suddetta missione un ulteriore mandato, quello di addestrare la guardia costiera e la marina libiche, con la speranza che magari, tra una decina d'anni, riusciranno loro negli obiettivi che EUNAVFOR Med ha sino ad oggi disatteso: mettere fuori uso le reti dei trafficanti. Ragion per cui o vi è l'impegno del Governo a sollecitare l'ONU e le autorità libiche affinché a breve si dia corso alla fase 3 della missione, permettendo quindi di entrare in acque libiche per impedire le partenze e contrastare il traffico di esseri umani, o viceversa si sospenda la missione, poiché le finalità per cui essa era nata sono state disattese. In questo caso, signor Sottosegretario, si riutilizzino le ingenti risorse impiegate per altri scopi più consoni alla sicurezza del Paese. Per esempio, si rafforzi, stavamo per dire, quella missione molto seria, denominata Mare sicuro, messa in campo dalla Difesa, opportunamente immaginata per scopi di sorveglianza e sicurezza del traffico marittimo, nonché per la tutela delle nostre piattaforme petrolifere, quindi dei nostri interessi energetici ed economici. economici. Sennonché, anche la missione Mare sicuro sembra risentire dell'onda emotiva e umanitaristica che avviluppa persino gli ammiragli che la comandano, i quali dalle pagine dei giornali comunicano tutta la loro commozione nell'eseguire i dovuti, peraltro, salvataggi in mare. Fiumi di retorica a gogò, se anche lo *speaker* della parata del 2 giugno scorso, nell'illustrare la missione, ha solamente ritenuto di ricordare che tale missione si è distinta per i numerosi salvataggi operati, tralasciando i reali obiettivi per cui è nata. Obiettivi primari e rilevantissimi, e se le navi della flotta vengono distolte dal loro compito principale, il dispositivo navale posto a garantire la sicurezza viene meno. Il che non vuol dire, naturalmente, che bisogna evitare i salvataggi; vuol dire, viceversa, che l'emergenza non può continuare all'infinito e che non è più possibile, con le varie operazioni messe in campo dai Governi di centrosinistra, lanciare continui messaggi incentivanti ai disperati di un intero Continente, che partono sapendo che, tanto, la Marina italiana li soccorrerà fin sotto le coste libiche. Non è con la nave Cavour che si fanno queste operazioni; semmai, con la nave Caronte delle Ferrovie dello Stato. Incentivare vuol dire, inoltre, contribuire alle tante morti che le traversate della speranza comportano. Per non parlare poi dei naturali rischi che l'immigrazione incontrollata determina in tema di sicurezza, rischi che non possono essere smentiti né dalle parole indelebilmente inutili del Ministro dell'interno, né dalle dichiarazioni ripetute di ammiragli e comandanti messi a capo delle missioni, i quali escludono sempre e comunque tale rischio, sposando le parole d'ordine del Governo. Una immigrazione poco governata, al contrario, costituisce un serissimo rischio per la sicurezza, che non può essere affrontato in modo leggero e distratto, se è vero che nulla si sa di decine dì migliaia di clandestini sbarcati negli ultimi anni sulle nostre coste, di cui si sono perse le tracce. Ad ogni modo, questo seguitare a cavalcare le emozioni per giustificare l'accoglienza a tutti i costi ha semplicemente favorito l'immigrazione clandestina senza avere minimamente scalfito le organizzazioni criminali che lucrano sul fenomeno. Ed è oltremodo risibile che il *Premier* si ostini a negare l'emergenza, preferendo insultare gli avversari politici che esprimono valutazioni diverse, arrivando persino a definirli meschini. Presidente, trovo invece meschino un *Premier* che utilizza, nei vari *talk show*, solo l'argomento degli stipendi dei senatori per giustificare la riforma del Senato. Ed è veramente sconcertante, per non dire che cadono le braccia, che un Primo Ministro ricorra al peggior populismo, adoperando argomenti non all'altezza di una riforma della Costituzione. Per tornare al nostro argomento, viceversa, l'emergenza esiste ed è sotto gli occhi di tutti, destinata ad acuirsi con la bella stagione in corso, e non sarà l'accoglienza a tutti i costi a risolvere questo epocale problema. Riteniamo invece necessario che il Governo si attrezzi, una volta per tutte, per tutelare e difendere i nostri confini, secondo i nostri interessi che prevedono comunque, in primo luogo, la celere e fondamentale stabilizzazione della Libia ed il conseguente controllo delle sue coste, oltre alla creazione di zone di extraterritorialità, dove poter esaminare chi ha diritto allo *status* di rifugiato e chi no. In questo senso servono anche accordi con la Tunisia e l'Egitto. Purtroppo, con quest'ultimo Paese il clima non è sereno per le note vicende e forse sarebbe il caso di chiedersi se il Governo italiano si sia mosso in maniera adeguata per avere la verità sul caso del giovane italiano assassinato. Da parte nostra, crediamo che la contrapposizione non solo possa allontanare la verità, ma compromettere anche i nostri interessi nazionali e strategici. Molti migranti, infatti, salpano dall'Egitto che, inoltre, in Libia sostiene il generale Haftar, osteggiato dal nostro Governo, nonostante fosse l'unico riconosciuto dalla Comunità internazionale, sino a ieri. Siamo il secondo *partner* commerciale dell'Egitto, dopo la Germania. Ci chiediamo, quindi, se il cancellare tutto questo, come qualcuno pretende, possa privarci della possibilità di richiedere con forza, ma senza spazientirci, la verità sul caso Regeni. Già il richiamo dell'ambasciatore sembrerebbe una forzatura, anche se gli egiziani sono stati poco collaborativi. Ma è un modo di fare, quello del Governo italiano, basato perlopiù su spinte emotive imposte dai *media*, che difficilmente consentirà di scoprire la verità su questo truce delitto. Un Governo serio, invece, la verità la pretende con forza lavorando a tutti i livelli, con la diplomazia ed anche sottobanco, salvaguardando ai tempo stesso i rapporti con un Paese alleato e i nostri interessi, evitando di sfruttare il dramma di una famiglia che ha perso un figlio in modo barbaro. Non giova, pertanto, far passare emendamenti che tendono ad esacerbare il clima, pur comprendendo il gesto simbolico dei proponenti nella richiesta di sospendere la consegna dei pezzi di ricambio degli aerei F-16, indebolendo in tal modo un Paese in lotta con il terrorismo. Non è con le misure simboliche, studiate magari per dare un contentino all'ala sinistra del PD, tifosa dei Fratelli Musulmani, che si faranno passi verso la verità sulla vicenda del ricercatore italiano. Abbiate allora il coraggio, signori del Governo, di ritirare l'ENI dall'Egitto, da Zara, dove è stato rinvenuto il più importante giacimento di gas. Pensare di piegare un regime militare con misure economiche demagogiche è cosa alquanto ridicola ed anche ipocrita. Per tornare alle missioni, questo Governo si è affannato nei mesi scorsi, rompendo i timpani a tutto il mondo, a rivendicare il comando di un coalizione internazionale per stabilizzare la Libia. Una brama di comando ed una smania risultati poi inutili, considerato che il neo costituito governo libico, non ritiene opportuno l'aiuto di una coalizione internazionale. Da qui la rinnovata ed apprezzata cautela del nostro Governo, principale sponsor del *premier* al-Sarraj, al quale si augura di accreditarsi presto presso il suo popolo, riuscendo nel contempo a combattere con successo il terrorismo insediatosi da quelle parti, cioè dietro l'uscio di casa nostra. È utile, comunque, ricordare che per noi il problema maggiore rimane l'immigrazione incontrollata e risulta decisivo in tempi brevi governare le coste libiche. bene la stabilizzazione della Libia, bene l'addestramento della Guardia costiera e della Marina libiche, ma senza aspettare all'infinito, impegnandosi celermente a sollecitare misure per impedire la partenza dei barconi e contrastare il traffico di esseri umani, avendo, in ogni caso, il nostro Paese le professionalità per smantellare le reti criminali che presiedono al turpe traffico. Si impegni in tal senso, quindi, il Governo italiano evitando che la cautela e la prudenza non si trasformino in colpevole letargo. *(Applausi

puntuale e anche una riaffermazione della nostra strategia di politica estera quale era - mi pare - largamente esplicitata nelle relazioni che abbiamo portato all'Assemblea. Le uniche cose che mi sento di sottolineare, per dare il quadro politico delle circostanze nelle quali operiamo, sono le seguenti: le missioni militari che stiamo per votare e approvare

nel tentativo di stabilizzare le aree di crisi del mondo e di intervenire a sostegno delle popolazioni che si trovano in una condizione di difficoltà. Non c'è nessun rituale nell'impegno di migliaia di nostri militari che ogni giorno riempiono d'orgoglio e dovrebbero riempire d'orgoglio il nostro Paese per l'azione che stanno facendo. Così come non è rituale il fatto che, anche con questo provvedimento, decidiamo di spostare una quota di militari a protezione della diga di Mossul a sostegno del contingente già presente e dell'azienda italiana che è chiamata a operare per consolidare quella infrastruttura. Se sono vere le proiezioni delle Nazioni Unite, in caso di un malaugurato crollo di quella diga o di un incidente sarebbero davvero centinaia di migliaia le vittime. Ma soprattutto si creerebbe una condizione di

siamo lì anche per affermare il fatto che quella diga, che è un prodotto dell'ingegneria e del talento italiano, è uno degli interventi che l'Italia fa all'estero dimostrando il proprio livello imprenditoriale, tecnologico e il proprio grande livello culturale. parte di questo intervento di natura imprenditoriale e tecnologico vede anche l'impegno dello Stato a sostegno delle imprese che intervengono e a sostegno di una grande

Così come credo che dobbiamo essere impegnati - l'abbiamo già detto più volte in questa sede - per la stabilizzazione della situazione in Libia. La situazione in Libia è in forte evoluzione.

questa stabilizzazione è necessaria e fondamentale per riuscire anche a far evolvere la nostra politica nel Mediterraneo e la politica verso i profughi che ci sono nel Mediterraneo. Devo dire che ho sentito cose curiose oggi, compreso il fatto che le persone che affondano sui barconi sarebbero i ricchi che vengono dall'Africa e che possono permettersi il viaggio. Cose che sarebbero curiose se non avessero in sé un profilo di di difficoltà a comprendere un processo che non è soltanto verso l'Italia e non coinvolge solo il nostro Paese ma è un processo globale che vede lo spostamento di interi popoli e che certamente non possiamo affrontare da soli, ma con una maggiore convergenza con l'Europa e le altre grandi potenze mondiali. La stabilizzazione della Libia è un fatto assolutamente fondamentale così come è fondamentale che vi sia il presidio del mare non per un doveroso salvataggio dei naufraghi - perché salvare i naufraghi è ciò che si deve fare quando ci sono dei naufraghi - bensì perché presidiare il Mediterraneo, avere i nostri contingenti militari a presidio del Mediterraneo, è ciò che si deve fare quando si vuole essere una potenza che vuole recitare un ruolo europeo e un ruolo mondiale. Abbiamo anche presentato un emendamento - simbolico è vero, lo voglio dire perché ne riparleremo - che riguarda la fornitura di ricambi per aeroplani all'Egitto. È - ripeto - un emendamento assolutamente simbolico,

la dolorosissima vicenda che ha visto anche quest'Assemblea impegnata a chiedere al Governo egiziano di fare chiarezza e di dare supporto

Certo che è una vicenda che ha profili oscuri ma non è una vicenda dalla quale facciamo derivare un mutamento di atteggiamento nei confronti dell'Egitto che sappiamo bene essere una potenza impegnata contro il terrorismo, un grande Paese arabo complesso, sappiamo bene essere un Paese che con noi ha molti collegamenti; e sappiamo bene che proprio in virtù dall'amicizia che ci ha legato a questo Paese noi abbiamo bisogno che su una vicenda come questa vi sia chiarezza. Dare un segnale simbolico forte è una cosa, dire che piuttosto sarebbe meglio rompere le relazioni economiche con l'Egitto è tutt'altro genere di considerazione e non era affatto nella nostra intenzione proporre corbellerie di questo tipo.

dentro la nostra politica estera c'è l'atteggiamento di un Paese che è un medio Paese mondiale ma che nella politica internazionale ricopre un ruolo di primo piano.

Nelle missioni militari c'è questa funzione. Anch'io sono dell'idea - sebbene non sia di mia competenza questo problema - che dovremmo affrontarlo, così come abbiamo fatto al Senato e alla Camera, con una legge quadro sulle missioni militari che ci consenta di definire con una programmazione stabile del Governo, il nostro impegno nell'intervento militare come parte della nostra politica estera. Questo è quello che dovremmo fare dall'anno prossimo ma già quest'anno

abbiamo sempre ribadito che il Governo è assolutamente favorevole e ha seguito fin dall'inizio la formulazione della legge quadro. In tal senso, continuiamo ad essere vicini a tutte le attività parlamentari relative alla legge quadro e, anche dell'attività di Governo, crediamo che sia assolutamente rilevante che la legge venga approvata il prima possibile. La seconda specifica riguarda la scopertura giuridica del personale militare,

alla risoluzione approvata ieri. Nel merito, il Governo si impegna affinché nelle sedi competenti (ONU e Governo libico), possa essere posto in essere, nel più breve tempo possibile, l'inizio della fase 3 della missione EUNAVFOR Med,

Il problema è che non abbiamo una situazione legislativa chiara, per cui tutto quello che è stato fatto è avviare un biomonitoraggio sugli abitanti. abitanti. Quindi milioni di persone ancora ignorano quali siano le loro condizioni. Si stanno facendo esami del sangue, ma milioni di veneti ignorano le loro condizioni.

ma, nel recepirla, abbiamo semplicemente detto che le Regioni dovranno rispettare gli *standard* di qualità ambientale entro il 2018. la direttiva del 2013 e abbiamo detto che entro il 2018 si dovranno rispettare gli *standard* di qualità: abbiamo deciso di non decidere, ma solo di rimandare.

e, alla fine, semplicemente ci fa morire. Siamo nella situazione classica in cui, per l'ennesima volta, anziché far valere nella pratica il principio di precauzione (non sono sicuro dei danni, quindi mi astengo dall'avvelenare),

Della serie "cornuti e mazziati"; non solo veniamo avvelenati, ma paghiamo anche: in questo momento sono i Comuni che pagano di tasca propria i filtri per tamponare la situazione. Quindi le aziende inquinano e noi paghiamo. In questo caso ci vorrebbe Totò, ma io non sono bravo In tutto questo il Ministero tace: i sindaci interessati alla situazione hanno chiesto indicazioni al Ministero della salute, ma finora non hanno ricevuto nessuna risposta in merito.

la beffa, che consiste nel fatto che ci dicono di non preoccuparci perché l'acqua inquinata non viene utilizzata per scopi alimentari, ma solo per irrigare.

di porre rimedio a una situazione che di fatto oggi impedisce a diverse Chiese e confessioni religiose di ottenere il riconoscimento dei propri ministri di culto. Con quella interrogazione si faceva presente che ad oggi i limiti posti da una interpretazione del Consiglio di Stato per la nomina dei ministri di culto rendeva e rende più difficile la conclusione dei percorsi in corso per la sottoscrizione di accordi e convenzioni tra Stato e confessioni religiose. Non solo, tutto ciò

rischiando di contraddire un diritto costituzionale fondamentale, come è appunto quello di poter praticare la propria fede per tutti i cittadini italiani. Più recentemente, il 12 aprile 2016 il Governo, in Commissione affari costituzionali, ha accolto un ordine del giorno che lo impegna a riconsiderare una riduzione dei limiti numerici di fedeli necessari per l'approvazione e il riconoscimento dei ministri di culto, tenendo conto dei diversi criteri di aggregazione delle confessioni religiose sui territori e in ogni caso a non porre questo limite minimo a 500, così come è adesso. tre anni il Parlamento, il Governo stesso e gran parte delle forze politiche si sono espressi per risolvere una situazione che sta producendo difficoltà all'esercizio dei culti per molte Chiese e sta mettendo in difficoltà la stessa possibilità di svolgere le funzioni di assistenza che sono proprie di tante Chiese. Non solo. Bisogna porre fine a una situazione che rischia di indebolire il necessario rapporto chiaro, regolato e trasparente tra Stato e alcune religioni. In questi mesi, anche dopo l'approvazione da parte del Governo dell'ordine del giorno, molti ministri di culto stanno presentando le richieste di riconoscimento. Signora Presidente, svolgo questo intervento perché le cose che ho riassunto velocemente riguardano temi importanti come quello della libertà religiosa,

il deliberato della Commissione affari costituzionali e gli atti di sindacato ispettivo proposti da gran parte del Parlamento trovino subito una loro concretizzazione. Credo sia ormai indifferibile e non più rinviabile arrivare ad una deliberazione da parte del Ministro dell'interno che metta in campo tutte le misure necessarie per restituire la possibilità per restituire la possibilità per tutte le Chiese e per tutti i culti rispettosi dei dettami costituzionali di chiedere il riconoscimento dei propri ministri di culto. Grazie

nel primo pomeriggio. Poi sono stati presentati emendamenti che devono avere il parere della Commissione bilancio; ci auguriamo che, per domattina, questi siano pervenuti. Sicuramente c'è un problema di raccordo con la Commissione bilancio perché questa non ostacoli il procedere dei lavori dell'Assemblea. Per quanto riguarda il senatore Marton, mi spiace molto che non sia stato presente. Abbiamo cercato di avvertirlo, ma evidentemente era impegnato. Domani, in sede di illustrazione degli emendamenti riguardanti il primo articolo, mi auguro possa recuperare il tempo con un intervento più ampio. Credo che così potremo cercare di "risarcirlo" e consentirgli di esprimere la sua posizione.